Il relatore, senatore Girotto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, adottato dal Governo al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, giunge in Aula dopo un approfondito esame presso la 10a Commissione, che, sin dall'inizio della legislatura, si è mostrata sempre attenta alle dinamiche relative al mercato energetico e ai conseguenti effetti per gli utenti. Voglio infatti ricordare la recente approvazione, il 22 luglio 2021, di una risoluzione piuttosto corposa sull'affare assegnato a gennaio 2020 sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti (Atto n. 397). È da moltissimo tempo che stiamo affrontando il tema in maniera strutturale, in particolare in questi ultimi mesi, in cui i prezzi, dopo la profonda discesa che ha caratterizzato il 2020, hanno visto una decisa impennata al rialzo determinata da una brusca accelerazione di tutti i costi delle materie prime, in conseguenza delle difficoltà occorse nelle filiere di approvvigionamento a causa della pandemia e delle alte quotazioni dei permessi di emissione di anidride carbonica, con variazioni che, nel giro di pochi mesi, hanno proiettato i prezzi delle materie prime decisamente verso massimi storici. L'incremento del costo dell'energia si è di recente ulteriormente acuito, con riferimento sia all'elettricità sia al gas. I forti aumenti sui prezzi dell'energia all'ingrosso hanno comportato un aumento delle tariffe elettriche di circa il 10 per cento nel terzo trimestre e di circa il 30 per cento nel quarto trimestre, aumenti peraltro limitati dall'intervento governativo (altrimenti sarebbero stati rispettivamente del 20 e del Tali aumenti, i più consistenti degli ultimi vent'anni, hanno portato ad un massimo storico del costo dell'energia elettrica per i consumatori. Gli interventi adottati dal Governo per complessivi 3,5 miliardi di euro, inclusa la riduzione dell'IVA sul gas, hanno consentito non solo di attenuare gli effetti degli aumenti del prezzo per l'energia elettrica e il gas naturale per 29 milioni di famiglie, oltre a 6 milioni di utenze elettriche non domestiche, in larghissima parte microimprese e piccole imprese, ma anche - e vorrei ricordarlo - di neutralizzare del tutto l'aumento dei prezzi per i titolari dei *bonus* sociali, cioè per le classi deboli, per chi è in situazione di difficoltà. Nel settore elettrico lo stanziamento, anche per il quarto trimestre 2021, di ulteriori risorse pari a 2 miliardi di euro, ha consentito all'Autorità di annullare completamente le aliquote degli oneri generali di sistema per tutti i clienti domestici e non domestici per altri usi, con potenza fino a 16,5 chilowatt, e di confermare il livello delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema, già praticamente dimezzato nel terzo trimestre 2021 per tutti gli altri utenti elettrici. Per la famiglia tipo l'annullamento degli oneri di sistema per il quarto trimestre 2021 ha avuto l'effetto di mitigare, di almeno il 12 per cento, la spesa totale per l'elettricità, che ha consentito di controbilanciare in parte l'aumento della componente relativa al prezzo dell'energia elettrica. Questo contesto, se da un lato sottolinea la vulnerabilità energetica del nostro Paese, che risente più degli altri Paesi europei della variazione dei prezzi delle *commodity*, con conseguente rischio di perdita di competitività dei nostri comparti *energy-intensive* e tensioni inflazionistiche destinate a deprimere i consumi, dall'altro mostra come l'incremento delle fonti rinnovabili, come previsto dal recente pacchetto climatico Fit for 55 e dal *green deal*, può avere un importante effetto benefico sull'economia del Paese. Secondo le analisi di Banca d'Italia, i rincari energetici possono comportare nel 2021 in media un aumento inferiore al 2 per cento dei costi complessivi delle imprese. Tuttavia l'impatto presenterà forti eterogeneità tra le imprese: per la maggior parte delle aziende l'aumento sarà modesto, ma potrebbe arrivare anche a tre volte il valore medio per quelle con una più elevata incidenza dei costi energetici. Il rialzo della bolletta energetica di imprese e famiglie avrà un impatto sull'inflazione al consumo, il cui aumento persisterà nei prossimi mesi, ma auspicabilmente non dovrebbe estendersi al medio termine. Ci tengo a ribadire che l'impatto dell'incremento dei costi energetici è stato contenuto grazie alla presenza di numerosi impianti da fonti rinnovabili nel sistema elettrico (abbiamo più di un milione di impianti da fonti rinnovabili), in particolare per le utenze domestiche e non domestiche che hanno autoprodotto l'energia che poi hanno consumato. Per tali aspetti ritengo sia urgente superare l'attuale modello energetico fossile, inquinante e centralizzato, garantendo la reale partecipazione e corretta concorrenza tra le diverse tecnologie che operano nel mercato elettrico. Ricordo che tale condizione non è ancora pienamente realizzata, poiché la mancanza di determinate norme tecniche rende, di fatto, tale mercato ancora centralizzato e alimentato prevalentemente da fonti fossili. E questo, cari colleghi, l'hanno capito in pochi. Mi spiace dirlo, ma l'hanno capito in pochissimi. Avremmo voluto tutti fare di più su questo provvedimento. Sono state presentate proposte emendative in numero contenuto ma significative, che avrebbero potuto contribuire a migliorare il testo e soprattutto a sostenere in maniera strutturale - quindi non *spot*, non sporadica - i cittadini utenti e le imprese: dall'estensione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, alla riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per ulteriori tipologie di utenti, agli interventi sugli oneri generali di sistema, alla concessione di garanzie da destinare alla realizzazione delle comunità energetiche, alla detrazione sulla realizzazione di accumuli, fino all'esenzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico con cavi e condutture per i venditori di energia elettrica e gas. Pur comprendendo che in questo momento le risorse necessarie risultano scarse o quasi nulle, visto l'approssimarsi dell'apertura della sessione di bilancio, non possiamo che auspicare che il Governo voglia tenere in considerazione la rilevanza delle misure proposte. Da molte Da molte di esse dipende realmente la transizione ecologica, la tutela dei soggetti vulnerabili, la riduzione della dipendenza energetica del Paese, il contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia, la crescita economica del Paese, la ricerca e l'innovazione tecnologica.

per tutte le utenze elettriche, di cui 700 milioni di euro specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Si tratta di somme dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, mentre gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021. In base al comma 2, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare per il quarto trimestre 2021 le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicati alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza fino a 16,5 kilowatt. A tale fine, entro il 15 dicembre 2021 sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro. L'articolo 2, comma 1, riduce l'aliquota IVA applicabile alla somministrazione di gas metano per usi civili e industriali. Il comma 2, al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, dispone che ARERA provveda a ridurre per il medesimo trimestre le aliquote relative agli oneri generali di gas, fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 15 dicembre 2021. L'articolo 3 assegna ad ARERA il compito di rideterminare per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate, aventi già diritto all'applicazione della tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica. L'articolo 4, al comma 1, reca l'abrogazione delle disposizioni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge e di contenuto variegato che, non avendo tempo, mi limito a elencare: elusione della razionalizzazione delle procedure contabili, valutazione ambientale preliminare, organici del personale amministrativo, istituti tecnici superiori, pubblica amministrazione con reclutamento e accesso e crediti acquisiti dagli ITS. L'articolo 4, comma 2, modifica la procedura con cui il corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria devono essere adeguate alle novità previste dall'articolo 12 12 della norma per l'accesso al corso di specializzazione. Il comma 3 dispone un'ulteriore proroga al 30 novembre 2021, in attesa di un apposito decreto, del termine per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica per evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. Nel corso dell'esame in Commissione sono stati approvati pochi emendamenti, che vedremo tra poco. La Commissione poi ha approvato modifiche di carattere formale al testo del decreto-legge attraverso le proposte emendative 1.100, tit. 1 e coord. 1. Ringrazio gli uffici della 10a Commissione per il prezioso contributo

Innanzitutto il Governo è intervenuto in modo tempestivo quando si sono cominciate ad avere le avvisaglie relative all'aumento sia dell'energia elettrica che del metano e ha stanziato una serie di risorse e - lo rifarà - abbiamo sentito in merito anche il Presidente del Consiglio - con la manovra di bilancio. Il provvedimento, come ha ricordato il relatore, mette sul piatto, per quanto riguarda il quarto trimestre,

Ciò che, però, a mio avviso, dovrebbe essere un momento di riflessione del Parlamento è il fatto che l'aumento complessivo dei prezzi delle materie prime e l'inflazione

a protestare semplicemente per una questione attinente a uno strumento di salute pubblica come il *green* *pass* o, se preferite, come giustamente dovrebbe essere chiamato, il certificato sanitario. Mi sono chiesta se è possibile che sia solamente questo il motivo che porta tanta rabbia in un momento in cui alla fine il Paese, pur con tutte le difficoltà che conosciamo, si è ripreso, ha affrontato la campagna di vaccinazione, ha risolto una serie di problemi e ha attivato una serie di procedimenti, compreso il fatto che stanno tangibilmente arrivando i flussi finanziari dall'Europa.

sta interessando tantissimi settori. È di ieri la notizia che il Ministero dell'agricoltura ha assunto una serie di iniziative proprio per il contenimento dei prezzi di beni di primissimo consumo (come ad esempio del latte).

debba essere analizzata più a fondo. In primo luogo per capire che evidentemente ha radici diverse e probabilmente sono di natura economica, ma in secondo luogo perché abbiamo il dovere di spiegare anche quello che sta facendo il Governo, che in quest'Aula, rispondendo ad alcune interrogazioni, ha confermato il fatto di avere la massima attenzione su queste tematiche, perché non c'è solo il problema contingente di questo aumento del prezzo del carburante e delle materie prime, ma c'è la necessità

aumenti sconsiderati di generi che definisco - tanto per capirci - di primo consumo, cioè quello che si fa normalmente. quindi da un lato il dovere di comprendere, ma dall'altro anche il dovere di spiegare il fatto che

e con forza il percorso che ci deve portare ad un'autonomia strategica, che vuol dire che se l'Europa - e con l'Europa l'Italia - dipende da troppi Paesi esteri per tutta una serie di forniture, è chiaro che poi si trova a dover combattere con l'inflazione da una parte, ma soprattutto con questo aumento dei prezzi, perché non riesce a governare il sistema.

le azioni che si stanno ponendo in essere per consentire la diversificazione degli approvvigionamenti delle materie prime. Il relatore ha ricordato un aspetto che condivido, per fare un esempio di come si possa reagire. Per molte famiglie, l'impatto relativo alle bollette elettriche è stato limitato

voglio dire che dobbiamo essere consapevoli che le azioni e soprattutto le risorse che il Governo stanzia per il problema delle bollette di energia elettrica e gas metano

per evitare una problematica legata a inflazione, aumento dei prezzi e altro ancora

rischiamo che i tanti sforzi che stiamo facendo adesso non vengano percepiti con la dovuta attenzione nel Paese, o magari si trasformino

acciaio, rame, minerali come il magnesio, alluminio, petrolio, metano

- la ripresa che timidamente un anno fa, dopo alcuni mesi di *lockdown*, il mondo globalizzato ha cominciato a intraprendere. Oggi famiglie e aziende

dà ancora segni di crescita. Atteso che gli analisti del mercato abbiano ragione nel dire che dopo il primo semestre del nuovo anno i prezzi torneranno a scendere, resterebbe comunque da passare un lungo inverno. chiaro anche che la crescita del costo dell'energia ha ripercussioni dirette su tutti i prodotti (dalle materie prime per l'estrazione, ai lavorati), ma anche sui servizi. Qualcuno ha parlato di concomitanza e tempesta perfetta. Io parlerei di addendi di semplici eventi che, sommati, hanno poi dato un gravoso totale. *in primis,* alla richiesta dei Paesi asiatici, che hanno ripreso a pieno ritmo la loro attività produttiva un po' prima dell'Europa, ma anche ai processi di trasformazione dei sistemi di combustione di tante acciaierie, da carbone a metano. Penso alla riduzione di produzione degli impianti eolici del Nord Europa, dovuta semplicemente ad aspetti di carattere climatico (i venti non ci sono stati). Penso inoltre alla riduzione dell'estrazione del metano in Norvegia per semplici interventi manutentivi che sono stati eseguiti durante il periodo del *lockdown*. Ci sono dunque tanti fattori e varie cause, che in un sistema economico come il nostro, diventato incontenibilmente energivoro, hanno generato l'ennesima pesante crisi. Onorevoli sono passati quasi cinquanta anni, ma tanti di noi si ricorderanno dell'*austerity*, quando il Consiglio dei ministri, convocato il 22 novembre 1973, varò diverse misure restrittive. La domenica si andava in giro con la bicicletta e confesso che da ragazzino ne ero anche felice. Fu vietata la circolazione dei mezzi motorizzati privati e i velivoli, fu ridotta la pubblica illuminazione delle città e i locali cominciarono a chiudere prima la sera. C'entrava anche allora il canale di Suez, che anche qualche mese fa è rimasto bloccato, sebbene per un breve periodo, un altro carico sul problema dell'incremento dei costi delle materie prime che oggi stiamo soffrendo. che allora non c'era la dipendenza che abbiamo oggi nell'uso dell'energia, ma continua a esserci la medesima dipendenza che avevamo allora nei confronti di materie prime che non possediamo, se non per esigue quantità: mi riferisco nella fattispecie proprio al metano e al petrolio. Con il provvedimento in esame, che cerca di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi, con una parziale compensazione di quelli che vengono definiti oneri generali di sistema per il trimestre in corso, con la riduzione dell'aliquota IVA e il rafforzamento del *bonus* sociale per i clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, è certo che andiamo a mettere una toppa ad uno spiffero freddo che entra in casa nostra e lo facciamo per la prima parte della stagione invernale.

però convinto del fatto che una quota residuale di tipo strutturale rimarrà comunque, perché epocali sono i fenomeni che stiamo vivendo in questo inoltrato inizio di secolo, epocale è il fenomeno pandemico globale, come è epocale il cambio di passo di tanti Paesi che stanno vivendo una nuova rivoluzione industriale, che sta cambiando le sorti del pianeta, e la sempre maggiore richiesta di materie prime, dai metalli, alle risorse agroalimentari, come accennavo in Tornando al tema delle risorse energetiche, oggi più che in passato occorre lavorare con urgenza ad un piano strategico nazionale *(Applausi)*, delle problematiche che sinteticamente ho testé riportato e della tanto conclamata e necessaria transizione sostenibile, compatibile con le esigenze di un sistema industriale in esercizio - non dimentichiamolo ma che soprattutto cerchi di colmare la dipendenza da materie prime, che sappiamo procurarci, ma che non abbiamo, per le quali siamo soggetti alle fluttuazioni del prezzo, secondo le classiche ed elementari leggi di mercato, della domanda e dell'offerta. Oggi la transizione eco-sostenibile potrebbe diventare per l'Italia perfino economicamente vantaggiosa. Mi spiego meglio: l'unica fonte di energia di cui il pianeta dispone è quella solare e da questa poi derivano il vento, l'acqua utilizzabile in termini di energia cinetica, le biomasse, ma anche il metano, il petrolio e il carbone. È certo che in Italia abbiamo il sole, il vento, l'acqua in centinaia di invasi già realizzati e costruiti, e anche le biomasse. Ebbene, è su queste fonti (sole, vento, acqua e biomasse) che dobbiamo lavorare e investire con urgenza, proprio per ridurre la dipendenza dal metano e dal petrolio. Abbiamo iniziato e dobbiamo continuare, accelerando i processi necessari; lo dobbiamo fare sfruttando tutte le risorse diffuse, anche le più piccole. Dobbiamo utilizzare i tetti di cui disponiamo, quelli degli edifici industriali, artigianali e civili; dobbiamo utilizzare il vento, il moto ondoso, gli invasi artificiali esistenti. Voglio puntualizzare anche un aspetto fondamentale: mi voglio soffermare sull'esigenza, non più procrastinabile, di riuscire a superare il limite dell'accumulo dell'energia elettrica. Mi riferisco al fatto che siamo spesso costretti a fermare gli impianti di produzione da fonte rinnovabile; forse non tutti siamo al corrente di questo fatto. Accade tante volte di dover bloccare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nei periodi in cui la richiesta dell'utenza è minima; ad esempio accade di dover fermare gli impianti eolici eolici esistenti. La soluzione c'è ed è quella di accumulare l'energia che si può già produrre e i cui picchi vengono tagliati. i cui picchi vengono tagliati. E lo possiamo fare nel modo più pulito e nel massimo rispetto dell'ambiente, raccogliendo il deflusso degli impianti idroelettrici in bacini a quota inferiore per ripomparlo, con l'energia dei picchi da fonte rinnovabile che oggi tagliamo, nell'invaso originario a quota superiore. Questi interventi non si fanno in pochi mesi, né in un anno; proprio per questo serve un piano urgente che programmi i necessari studi di fattibilità. Diversamente, rincorreremo sempre in emergenza, con provvedimenti urgenti. Oggi è il momento di programmare, nel rispetto del nostro pianeta; i fondi ci sono. È una richiesta espressa che avanzo al Governo.

capita raramente, nella storia di un Paese, che un decreto-legge così breve e così piccolo (appena tre articoli che parlano di bollette, più altri tre che parlano di altro) abbia una ricaduta così ampia sulla popolazione. In tre articoli praticamente ci prendiamo cura di tutte le famiglie italiane e di una parte importante delle piccole e piccolissime imprese. Lo facciamo ovviamente a tempo limitato, fino a dicembre, a dicembre, per attenuare un momento di disagio, che però - com'è stato ampiamente descritto in quest'Aula - è un disagio di lungo periodo, periodo, che proviene non dall'Italia, ma dai venti freddi dell'Europa dell'est e che ha origini lontane.

è proprio la nostra incapacità di programmare una politica energetica per tempo. Non è un caso che il vice presidente della Commissione europea Timmermans abbia quasi chiesto scusa ai cittadini europei, dicendo avessimo iniziato dieci anni prima le politiche sulle energie rinnovabili, oggi non ci saremmo trovati in questa condizione. Il mio intervento si concentrerà sui primi tre articoli di questo decreto-legge, perché l'articolo 4 parla totalmente di altro, con buona pace di chi, dal Colle in giù, dice che i decreti-legge devono essere omogenei.

concentrarsi sul nostro orizzonte temporale futuro, ovvero verso le energie rinnovabili, verso una sostenibilità energetica migliore. Ovviamente questo è avvenuto con gli ultimi due Governi, Conte 1 e Conte 2; prima si è fatto veramente ben poco.

da usi impropri a usi propri e rivoluzionari, si creano milioni di posti di lavoro. Solo il superbonus ha creato 135.000 unità di lavoro in più. Signori, sono dati reali; sono persone occupate, imprese che stanno lavorando e che porteranno nel lungo periodo l'effetto di ridurre l'uso dei fossili, e se riduciamo l'uso dei fossili, ridurremo anche la bolletta energetica perché le bollette energetiche riflettono semplicemente la più vecchia legge dell'economia, la legge della domanda e dell'offerta: riduci la domanda di energia, abbassi il costo dell'energia. Ecco che con una legge che abbiamo indirizzato al settore civile, che è responsabile dell'uso del 40 per cento dell'energia, ci ritroviamo con maggiore resistenza e resilienza del nostro sistema

le varie sollecitazioni che provengono da tutto il mondo imprenditoriale: Confindustria, imprese, banche, tutto il mondo che, grazie a questa legge, si è messo in moto.

che poi rivendono il gas sui mercati internazionali; quindi, potremmo anche raddoppiare la produzione e non arrivare sostanzialmente ad alcun risultato. Non serve a niente trivellare maggiormente

Per far capire un po' quello di cui stiamo parlando. Tutto questo ci spinge verso un uso più responsabile e migliore dell'energia. Dobbiamo ridurre l'uso del gas. Se vogliamo abbassare il costo delle bollette agli italiani, dobbiamo diminuire gli usi del gas e non aumentarne la produzione. Questa è la logica dell'idraulico: se hai una perdita, vai a riparare il danno e non ad

il costo delle bollette agli italiani - udite, udite - usando i soldi del reddito di cittadinanza. Questa è veramente bellissima. Mi sono messo a ridere per non piangere:

è stato dimostrato essere inutile, antieconomica e contro l'ambiente. E adesso noi vogliamo implementarla in Italia? No, noi dobbiamo attuare l'unica misura possibile per catturare e sequestrare la CO2 e cioè piantare più alberi. Dobbiamo piantare miliardi di alberi, come è stato stabilito nella

tutti gli emendamenti che per mancanza di copertura sono stati bocciati e vado anche qui a favore dei venditori di energia elettrica e gas che pagano in più oneri concessori ai Comuni, riversando

Signor Presidente, al di là dei toni trionfalistici che abbiamo appena ascoltato e delle dichiarazioni ed enunciazioni

tutto sia emergenza anche quando ormai la pandemia o i problemi energetici sono di dominio pubblico da anni, ci si rende conto e si viene ogni volta travolti dalle emergenze come se fossero processi ineludibili e assolutamente non preventivabili o quanto meno non pianificabili. Credo invece che ci sia un problema di base. Manca una strategia energetica, problema acuito, tra l'altro, da una visione prettamente ideologica di quella che dovrebbe essere la transizione ecologica, cioè di quella che dovrebbe essere l'energia non oggi ma tra qualche anno. Al Al di là di questo, sono convinto tra l'altro che la continua decretazione di emergenza e il continuo rincorrere le questioni non aiutino nemmeno la fiducia che i cittadini poi hanno nei confronti di questo Parlamento e anche di questo Governo. Ipotizziamo che sia vero che c'è stato un effetto Draghi,

Faccio il sindaco e nel mio Comune - come in tutti gli 8.000 Comuni d'Italia - quando c'è un problema, quando c'è un'emergenza, è atavico che, indipendentemente dal colore del sindaco, la popolazione si stringa attorno a lui e lo veda come punto di riferimento; è una cosa pressoché normale. È accaduta la stessa cosa con Draghi. Oggi però tanti nodi stanno venendo al pettine, soprattutto grazie al fatto che ci si trova nel semestre bianco e quindi i partiti politici che sostengono la maggioranza, che fino a ieri in qualche maniera piegavano il capo oppure, con una forma di accondiscendenza un po' forzata, non osavano nemmeno criticare l'operato di Draghi, abbiamo visto che invece cominciano ad alzare un po' la una volta votato il Presidente della Repubblica, ci si liberi anche di quello che ormai cominciano a definire "il fardello Draghi", per riprendere un controllo un po' più preciso e puntuale

altre. In Portogallo infatti di questi aumenti dell'energia non se n'è accorto nessuno; in Francia se ne sono accorti in maniera - diciamo così - leggera; in Italia, guarda caso, i cittadini se ne accorgono dalle bollette. Addirittura vi è un Governo che annuncia l'aumento delle bollette e che, anziché pianificare da subito un intervento, prima si premura di mettere la mano avanti dicendo che aumenteranno le bollette e dopo, quasi con una missione salvifica,

Babbo Natale), riuscendo quasi a farci credere che se non ci fosse stato questo Governo oggi, le bollette sarebbero esponenzialmente più alte. Mi sembra leggermente disonesto intellettualmente il solo pensare che possa essere così. In realtà, quello che è accaduto è molto più semplice: manca una strategia nazionale sull'energia; molto più probabilmente, manca una vera strategia nazionale che vada al di là del contingente. Non c'è un Governo di lunga veduta e non può esserci, perché questa è una maggioranza raffazzonata che va dalla Lega e Forza Italia al MoVimento 5 Stelle, e che non può avere una visione strategica della Nazione, essa ci sono dentro almeno cinque visioni differenti della Nazione. È evidente che continuate sempre ad arrovellarvi sulla vostra presunta capacità di risolvere i problemi attuali. In realtà, i problemi oggi non è che vengono solo dalle bollette delle famiglie.

che, se non esiste una politica di pianificazione, non si accontenta di sapere che dal 2023 - come voi dite - le bollette torneranno al valore del 2020. del 2020. Per quanto voi possiate essere credibili, non credo che la maggior parte degli italiani creda alle vostre favole; nella stessa maniera non ci credono perché lo toccano con mano tutti i giorni e si rendono conto che non è possibile per loro affrontare almeno un anno e mezzo in condizione di forte difficoltà. Sono costi e aumenti che non riguardano solo il settore artigianale. Pensiamo all'agricoltura, oggi si crede che la speculazione sui prezzi agricoli sia colpa degli agricoltori, ma in proposito ci sono sempre due visioni: quando si abbassano i prezzi non è merito degli agricoltori, ma della grande distribuzione e di chi sta sopra gli agricoltori; quando invece aumenta il costo delle materie prime è sempre colpa degli agricoltori, che, guarda caso, sono schiacciati dalla filiera e si vedono vedono riconoscere una legge sulle pratiche sleali che di fatto è una cartina tornasole, perché non risolve il loro grande problema della fissazione di un prezzo minimo, come già accadeva. In Italia avevamo l'ammasso del grano, lo abbiamo smantellato insieme ai grandi consorzi, convinti che lì si annidassero i costi della politica nazionale; poi ci siamo resi conto, invece, che il grande costo di questa Nazione è il non fare strategia e l'essere al traino della strategia altrui,

di questa mazzata che voi intendete dare al fato avverso, cioè all'aumento dei prezzi, si aggiunge quella da voi scelta, cioè di fare in modo che le imprese non trovino dipendenti, perché voi li pagate per rimanere a casa a non fare nulla. Non è quindi vero che siete a fianco delle imprese. Voi acuite la loro crisi con le vostre scelte

«prenditori», quindi quelli non si toccano. Visto che questi sono i preludi e questa è la situazione attuale, mi sembra evidente che noi siamo l'unico spicchio di Parlamento che oggi può addirittura

un grande impatto mediatico, come abbiamo registrato tutti quanti, la notizia che con le riaperture, il riavvio delle attività economiche e la ripresa

che ha avuto un grande impatto politico, però finalmente ha riportato al centro del dibattito politico stesso il tema del caro bollette. Da subito ci siamo mobilitati tutti quanti, le forze politiche e il Governo, perché una tegola di questo genere, in un momento così particolare per il nostro Paese, non doveva e non non deve esserci assolutamente. Siamo usciti da una fase difficile, finalmente intravediamo la luce in fondo al *tunnel,* quindi in questo momento particolare non possiamo assolutamente piegare i cittadini e le imprese con questi aumenti spropositati. Il tema del caro bollette è dunque ritornato prepotentemente al centro del dibattito politico,

di ridurre la produzione e i consumi di energia in questo momento particolare. Non ce lo possiamo permettere, perché nel momento in cui stiamo rincorrendo con forza la crescita del nostro Paese, non possiamo pensare che le aziende rallentino o sospendano persino la produzione. È una spirale pericolosa che va disinnescata,

e altri 20 milioni di clienti domestici per i quali vengono azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021.

gli effetti previsti dall'aumento della bolletta nel quarto trimestre 2021. Anche l'IVA sugli utenti di gas naturale, famiglie e imprese, che in molti casi è del 10 o del 22 per cento, è portata al 5 per cento e gli oneri di sistema sono azzerati. È una misura

che in questo momento particolare il Governo ha varato, proprio per far sentire, con forza, l'aiuto e il sostegno dello Stato nei confronti delle famiglie e delle imprese.

il tema della discussione odierna è quanto mai importante e vitale per tante famiglie ed aziende del nostro Paese. L'aumento incontrollato dei costi energetici rischia, infatti, di avere un impatto devastante sui bilanci, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, direttamente ed indirettamente. Direttamente, perché con la stagione invernale alle porte i consumi per luce e riscaldamento sono destinati a crescere; indirettamente, perché l'aumento dei costi energetici per le aziende, a cascata, provocherà un aumento di prezzi dei prodotti finiti, con il risultato di impattare ulteriormente in maniera negativa sui bilanci familiari, anche solo a livello dei costi da sostenere per fare la spesa, considerata la crescita combinata e finora incontrollata dei costi alla pompa del carburante. Basta vedere, già rispetto ad un anno fa, quanto siano aumentati i prezzi al dettaglio di molti prodotti. La situazione si è aggravata dopo che il costo dell'energia elettrica ha subito un deciso incremento dal secondo trimestre del 2020 all'agosto di quest'anno, passando da 16,08 a 22,89 centesimi di euro per kilowattora, stando ai prezzi del servizio di maggior tutela. Nel frattempo, però, i prezzi sono materialmente cresciuti in maniera considerevole. Basti pensare che il prezzo del petrolio è aumentato del 200 per cento dalla primavera del 2020 e quello del gas naturale del 30 per cento solo negli ultimi tre mesi. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante per la situazione del nostro Paese, visto che il gas naturale è impiegato per produrre il 40 per cento dell'energia elettrica. è stata provocata da una combinazione di fattori, tra i quali la minore disponibilità di gas prodotto direttamente in Europa e la diminuzione delle forniture dalla Russia, dalla quale l'Europa è fortemente dipendente in materia energetica. Senza volersi addentrare in considerazioni di ordine geopolitico, è evidente che la posizione dell'Italia è quanto mai debole, stando la notoria dipendenza energetica dalle forniture estere per coprire il fabbisogno interno. una condizione che in casi come questo, di aumento sconsiderato dei prezzi per effetto anche di indubbie speculazioni, accentua la fragilità della nostra economia. In tal senso, l'abbandono frettoloso della produzione energetica tramite centrali nucleari si sta rivelando dannoso per il nostro Paese dal punto di vista economico. Il tema delle energie rinnovabili è sfruttato sempre in maniera ideologica senza dati concreti, ma la verità è che circa il 10 per cento del consumo di energia elettrica in Italia deriva deriva dal nucleare ed è tutta di importazione, prevalentemente dalla vicina Francia, la quale peraltro produce circa il 75 per cento della propria energia elettrica con le centrali nucleari. nucleari. Noi abbiamo rinunciato a produrre energia nucleare per ragioni ambientali, ma la compriamo oltralpe, con il risultato che paghiamo qualcosa che avremmo potuto produrre in casa, senza per questo essere al riparo dai presunti rischi legati alla sua produzione. Se c'è una lezione che ci deve servire per la crisi in cui stiamo dibattendoci, questa è rappresentata dal fatto che dobbiamo lavorare per ridurre il più possibile la dipendenza dalle importazioni di energia. Se questo deve passare dalla reintroduzione di una produzione nucleare sfruttando le nuove tecnologie ad alta sicurezza e a basso impatto ambientale, allora è bene affrontare il tema, senza piegarsi alla propaganda strumentale dei fanatici dell'ambientalismo che, come ha detto qualcuno, provocano più danni della catastrofe climatica di cui si dibatte. Il Governo, con il provvedimento di cui discutiamo oggi, ha messo in campo misure straordinarie per attenuare gli effetti dell'impennata dei prezzi di gas e luce, impegnando complessivamente molte risorse. cifre imponenti, ma nemmeno lontanamente sufficienti per coprire l'aumento dei prezzi dell'energia che acquistiamo dall'estero. Infatti, con il pesante sforzo economico studiato dal Governo gli aumenti previsti in bolletta saranno del 29,08 per cento per la luce e del 14,04 per il gas, impattando comunque in maniera gravosa sui bilanci di tante famiglie, ma non solo. infatti, all'aumento dei costi delle altre materie prime come, ad esempio, l'acciaio e, combinandoli con gli aumenti del costo dell'energia, il risultato sarà di aumenti esorbitanti per i prodotti finali. Se il costo di produzione di un auto aumenta di pari passo con quello delle sue componenti, soprattutto delle parti in plastica e in acciaio, lo stesso avverrà in misura proporzionale con il prezzo al consumatore, con il risultato di diminuire la fetta di potenziali acquirenti. di auto si traduce in minor produzione e in minor lavoro *in primis* per gli operai delle fabbriche di assemblaggio e in seguito per le aziende della componentistica, in un circolo vizioso che potrebbe avere effetti drammatici sull'economia del nostro Paese. L'esempio del settore automobilistico potrebbe essere replicato anche per altri settori. L'incubo di una nuova brutta stagione non è così distante e ovviamente non riguarda solo il nostro Paese, ma l'intera Europa con le debite proporzioni. In questo momento le nostre aziende - parlo in particolare della mia zona, il Canavese, dove peraltro si stampa il 70 per cento dell'acciaio in Italia - stanno vivendo una fase di ripresa, dopo una stagnazione dovuta all'esplodere della pandemia. Questa fase, però, rischia di terminare ben presto se non si pone un freno alla spirale dell'aumento dei prezzi delle materie prime. In questo senso, l'Unione europea è chiamata a svolgere un ruolo straordinariamente importante per evitare, o almeno attenuare, gli effetti di una crisi economica dalle proporzioni ancora non ben definite in tutta la loro gravità. È evidente che l'Italia non può continuare all'infinito a immettere risorse per calmierare i costi dell'energia, serve una risposta strutturale per affrontare le sfide che la situazione attuale ci impone e per pianificare una strategia volta a metterci al riparo dalle dipendenze e dalle importazioni di risorse energetiche. Queste risposte non possono che venire dall'Europa, dove crediamo che il nostro Paese potrà tornare a recitare un ruolo di prim'ordine grazie anche all'autorevolezza, alla competenza e all'esperienza del nostro Presidente del Consiglio. Riguardo alle misure del giorno per contenere gli aumenti delle bollette energetiche, noi della Lega siamo sicuramente favorevoli, pur consapevoli del fatto che si tratta di un palliativo che non può risolvere da solo il problema. *(Applausi)*.

per le continue politiche energetiche intraprese da questo Paese nel passato che non sono all'altezza di quanto dobbiamo fare. Davanti a una transizione ecologica necessaria nel nostro Paese, richiesta dai giovani e dai movimenti come Fridays for Future, dall'azione di Greta Thunberg, richiesti dal nostro Pianeta e dagli sconvolgimenti climatici che tutte le città del nostro Paese vivono ormai da troppi anni, dovuti al surriscaldamento climatico per via delle emissioni dei gas serra, del metano, del CO2, direttamente responsabili, ci troviamo a dover trovare risorse per abbassare il costo dell'energia che consumiamo tutti i giorni. Ma perché ci troviamo a discutere di un provvedimento come questo? Per quale motivo dobbiamo ancora dipendere dai fossili in questo Paese? Per quale motivo continuiamo a parlare di CCS? Per quale motivo, in quest'Aula, continuiamo, dopo due *referendum*, a parlare di nucleare?

che hanno avuto vita grazie al lavoro del presidente Girotto e del sottosegretario Fraccaro. Siamo contenti che adesso tutti quanti parliate di super bonus, ma un anno e mezzo fa eravamo da soli a portare avanti questa tematica all'interno di quest'Assemblea. Adesso siamo tutti d'accordo che è necessario, manca la componente del Governo che capisca quanto è importante questo provvedimento. Dipendiamo da altri perché la politica

Il MoVimento 5 Stelle è stato la prima forza politica alla Camera, con Davide Crippa, a parlare del tema con una mozione contro il caro bollette,

Si interviene per cercare di fermare questi tariffari. Limitare i maxi rincari servirà ad aiutare le famiglie e le piccole imprese e a salvaguardare il nostro tessuto economico-sociale,

Ciò dimostra ancora una volta l'assoluta necessità di uscire dalla dipendenza dai fossili. Bisogna intervenire sulla crescita delle energie rinnovabili, sull'efficientamento energetico e sulla diffusione del sistema di accumulo. Logiche esterne all'Italia hanno portato le materie prime a dei massimi storici, a causa della pandemia, delle difficoltà delle filiere di approvvigionamento e delle alte quotazioni per i permessi di

Il provvedimento in esame nasce per contenere gli aumenti dei prezzi di gas ed energia elettrica nel quarto trimestre per circa 3 milioni di famiglie che beneficeranno di un *bonus* sociale elettrico, per i nuclei familiari numerosi,

Concludo con una dichiarazione del nostro presidente Conte proprio su questo tema. Sulla questione bollette il momento è propizio per una soluzione definitiva: dobbiamo cogliere l'occasione per alleggerire le bollette una volta per tutte, spostando gli oneri di sistema finalizzati agli investimenti di fonti rinnovabili e allo smantellamento del nucleare nella fiscalità generale, affinché vengano pagati in maniera proporzionale alla capacità di reddito personale, nel pieno rispetto del principio costituzionale della progressività dell'imposizione fiscale. Non ci vuole tanto per capire qual è la strada da intraprendere in questo momento. Il MoVimento 5 Stelle l'ha tracciata: comunità energetiche, *super bonus*, avvento della mobilità elettrica e incentivi

di cose che diciamo dal 2013. Stiamo infatti pagando le scelte sbagliate dei decenni passati e il Covid ha semplicemente portato i nodi al pettine. Non c'è molto altro da aggiungere: abbiamo sbagliato le politiche energetiche negli ultimi vent'anni. 2008-2009, con i costi di allora, che erano cinque volte superiori a quelli di adesso e con una efficienza che era comunque più o meno la metà di quella attuale, installammo 9 *gigawatt* di fotovoltaico.

tutte le centrali a gas che abbiamo realizzato negli ultimi vent'anni. Lo abbiamo fatto in un anno solo e con prezzi che erano cinque volte superiori a quelli attuali (scansando per un attimo l'aumento dovuto alla pandemia, che rientrerà). Quindi, a livello di rapporto tra costi e benefici, mi dispiace disilludere chi è convinto di poter perseguire altre strade, ma vinceranno le rinnovabili, semplicemente perché costano di meno. La California e la Florida, che non sono propriamente due Paesi governati dal MoVimento 5 Stelle o da associazioni ambientaliste - tra l'altro una è democratica e l'altra è repubblicana e quindi c'è la *par condicio* anche in questo caso stanno costruendo non centrali a gas, né tantomeno centrali nucleari, ma centrali a fonti rinnovabili, con affiancati gli stoccaggi, e lo fanno perché costa di meno. Quindi, se vogliamo passare ai fatti, dalle tante parole e dal "bla bla bla" che ho sentito anche oggi, dobbiamo fare una cosa molto semplice: aumentare la produzione delle rinnovabili e questo passa per una semplificazione delle procedure amministrative. Adesso vedremo

sia dal lato del superbonus. I colleghi hanno detto che con il superbonus tagliamo moltissimo i costi di fabbisogno energetico, ma ne approfitto, visto che ne ho facoltà, per dire che così tagliamo anche i costi sanitari.

non so chi di voi conosca il mercato del giorno prima, il mercato dei servizi di dispacciamento, il mercato dei servizi ancillari, gli aggregatori, il *capacity market*, ma se non riformeremo queste cose, chi sarà nuovamente nella prossima legislatura dovrà spiegare agli italiani perché in questa legislatura non abbiamo riformato il mercato elettrico, con la conseguenza di non essere pronti ad accogliere tutta la produzione da rinnovabili. a studiare di più questo argomento, perché altrimenti la transizione ecologica non si fa. La transizione ecologica per l'80 per cento è transizione energetica e la transizione energetica sono le rinnovabili; se il mercato elettrico non è pronto a recepire le rinnovabili, siamo punto e a capo. Qualcuno ha parlato del solito dibattito sull'aumento delle trivellazioni interne. A parte il fatto che il PiTESAI è molto restrittivo in questo senso

C'è sempre il discorso del prezzo: infatti gli investitori stanno venendo per installare le rinnovabili, non per fare nuovi pozzi di petrolio o di gas. Due parole anche sul nucleare, il famoso nucleare. nucleare. Do una notizia che evidentemente molti non sanno, semplicemente perché non è la loro materia; non gliene faccio una colpa, evidentemente sono esperti di altro. Vi faccio presente che questo famoso nucleare pulito ed economico, cioè la quarta generazione,

È come parlare della fusione nucleare: è una bellissima cosa, ma è ancora allo stadio prototipale. La quarta generazione potrebbe anche essere una bella cosa, ma non è stata assolutamente realizzata. Non parliamo poi dei costi, di cui nessuno ha idea. Anche a livello di sperimentazione e di prototipo, la quarta generazione, cioè una centrale fissile, non a fusione ma a fissione nucleare (pulita, sicura ed economica), non esiste; state parlando di una cosa che proprio non esiste. Leggete i testi scientifici: sono vent'anni che si parla di quarta generazione, ma non riusciamo nemmeno a fare la terza generazione, colleghi.

Colleghi, perché il nucleare va avanti? Togliamo la foglia di fico: il nucleare va avanti per questioni militari, esclusivamente per questioni militari. Sono i cittadini francesi che stanno pagando il nucleare. Vi do una notizia: Areva è fallita.

il mondo, non solo in Italia, non esiste un deposito di rifiuti nucleari della terza categoria, cioè quelli che durano 200.000 anni. Avete idea di cosa significa costruire un deposito che duri 200.000 anni? In che lingua scriviamo le istruzioni per un deposito che deve durare 200.000 anni? Su che supporto le mettiamo? Su carta, su DVD, su una schedina SD, su un computer, su un disco rigido?

passiamo alle riforme strutturali. Le riforme strutturali sono: più generazione distribuita, più rinnovabili, più efficienza energetica, superbonus, comunità energetiche. E buon lavoro a tutti.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 2.0.2.

però le voglio far notare che il titolo del decreto-legge arrivato all'attenzione del Senato e della Commissione reca: «Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento

perché c'è un comma che parla di modifiche dei piani di studio e di modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica? *(Applausi)*. Me lo sa spiegare, Presidente? Cosa c'entrano l'inclusione scolastica e i corsi di pedagogia con le bollette del gas?

lo stesso Governo e il Senato impediscono ai parlamentari di introdurre argomenti molto più attinenti, perché cade la tagliola dell'inammissibilità.

"nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi". Detto nel *latinorum* dei giuristi, significa che abbiamo messo una pezza giuridica al fatto che il decreto-legge contiene materie estranee al titolo dello stesso, però su questo nessuno dice niente, perché va tutto bene, se lo fa la maggioranza. Dopodiché,

chiamatela come volete, ma non è più tale. Mi rifaccio agli appelli che in anni recenti e meno recenti le massime autorità dello Stato hanno rivolto al Governo e al Parlamento in tema di decreti-legge *omnibus* so che non interessa ai colleghi, ma vorrei concludere. Mi rifaccio agli appelli istituzionali e accademici di chi, molto più preparato di me, ancora una volta ha denunciato il fatto che approviamo decreti *omnibus* senza alcun rispetto della Costituzione, del Parlamento, del Senato e delle forze di opposizione. Senatore Ciriani, la Presidenza ha tenuto in considerazione tempistiche che rendono la la norma non più temporale. Chiedo al senatore Girotto, che insieme alla presidente Alberti Casellati ha stabilito i termini per i quali l'emendamento è stato dichiarato improponibile, se vuole aggiungere riferimenti al senatore Ciriani per comprenderne l'improponibilità; altrimenti, come ben sa, essendo il giudizio della Presidenza inappellabile, considero l'emendamento improponibile, così come mi è stato indicato (per un problema di

Chiedo pertanto il ritiro dell'ordine del giorno G1.4 e la riammissione alla trattazione dell'ordine del giorno G2.16. un equivoco nella diversa numerazione degli ordini del giorno tra la Commissione e

Il primo è il G2.7 (testo 2), attraverso il quale chiediamo al Governo di utilizzare le risorse stanziate in legge di bilancio, a cui auspichiamo se ne possano aggiungere altre, per fare un intervento di mitigazione del caro energia per il primo trimestre

per ricomprendere anche le medie e le grandi imprese, gli energivori del gas, e anche - perché non sono esenti da questa batosta del caro energia - le amministrazioni comunali, che da qualche mese a questa parte hanno difficoltà a far quadrare i bilanci. chiediamo al Governo di valutare nel prossimo provvedimento che l'IVA agevolata sia erogata non solo alla somministrazione del gas, ma anche a quella

Presidente, vorrei chiedere se il relatore può illustrare meglio l'emendamento 4.5 (testo 2 corretto) della Commissione, perché non ho udito una sola parola di spiegazione, ma vorrei capirne bene il senso e il merito, se possibile. Mi è parsa un'illustrazione molto sbrigativa, quindi vorrei capire meglio i motivi, i contenuti e le finalità dell'emendamento - se è ancora possibile nel Parlamento fare una discussione tra maggioranza e opposizione - dato che il senatore Girotto non ne ha parlato affatto.

per provvedimenti che probabilmente neanche conosce né condivide, però, Presidente, ancora una volta facendo non solo opera di testimonianza, ma rendendo anche valore all'attività di questo Parlamento, che si è ridotto ad essere totalmente subalterno alle volontà del Governo qui approviamo commi e articoli che neanche il relatore conosce: non so se ci rendiamo conto della gravità della situazione. *(Commenti).* Il relatore ci ha appena detto che l'emendamento è autoesplicativo. Ancora una volta, ribadisco

dov'è l'urgenza di un comma inserito all'interno di un decreto-legge che riguarda le bollette energetiche, con valenza a decorrere dal 2025? Qualcuno me lo dovrà anche spiegare, prima o poi. So che siamo fastidiosi, perché ricordiamo all'Assemblea, ai colleghi e ai Gruppi che il Parlamento dovrebbe avere un minimo di dignità. Non si capisce perché è vietato al Parlamento

Qualcuno avrà un sussulto di dignità per bocciare questo comma e rimandarlo nella Commissione competente, che non è quella dell'energia, per valutarlo e presentarlo insieme con calma nel primo provvedimento utile e coerente? Possiamo fare questo lavoro o non è possibile?

la maggioranza non è in grado di spiegarci il contenuto dei testi.

Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, intervengo brevemente su questo testo. Sappiamo che il rincaro delle bollette di luce e gas era stato annunciato da tempo destato enorme preoccupazione, soprattutto in chi vive in condizioni di indigenza, dovute sia alla situazione personale, sia alle conseguenze della pandemia.

le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2 porteranno in tempi brevi a un aumento molto significativo, come ci è stato spiegato in maniera inequivocabile. Siamo anche in presenza di un incremento del costo delle materie prime più ampio ed imprevedibile rispetto ai precedenti. L'intervento celere e tempestivo del Governo - in questo senso, dobbiamo un ringraziamento, ancora una volta, all'attenzione e alla solerzia dell'Esecutivo verso queste patologie e criticità criticità - che è confluito in questo decreto-legge cerca quindi di ammorbidirne gli effetti in una fase delicata della ripresa per proteggere i consumatori più fragili e più esposti.

in quanto quello stato di indigenza, come sappiamo, ha raggiunto anche una percentuale di famiglie e di imprese che, pur essendo nella media, ormai faticano a sopportare la quotidianità. A maggior ragione, quindi, è necessario un lavoro per sfruttare tutte le opportunità di riduzione strutturale dei costi energetici e in questa direzione si è mossa anche la 10a Commissione, a cui va evidentemente un ringraziamento da parte di tutti noi per il lavoro svolto, nei margini di ciò che era possibile fare, cercando di migliorare il testo originale. Penso anche a un emendamento che è stato fortemente voluto dal Gruppo Italia Viva - Partito Socialista Italiano, che predispone misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e contestualmente ridurre quindi i costi delle transizioni. Il rincaro delle bollette costituisce indubbiamente l'ennesimo problema, l'ennesima criticità che si somma all'impoverimento generale dovuto alla crisi economica, da quando è esplosa la pandemia ai giorni nostri. È una situazione che non riguarda solo una piccola parte del Paese, ma travolge in maniera trasversale molte famiglie, molte imprese e anche molti giovani, che si trovano a fare i conti con le spese connesse alla necessità di mantenersi autonomamente, a fronte però di un lavoro il più delle volte precario, a tempo determinato, che non garantisce stabilità e serenità nella conduzione della quotidianità. In questo quadro, quindi, l'intervento del Governo si è rivelato assolutamente indispensabile e necessario. Ancora una volta, è chiara la testimonianza del fatto che il Governo ha saputo e continua a intercettare tutte le difficoltà che il Paese sta vivendo e ha predisposto un provvedimento che sarà in grado non certamente di risolvere, ma almeno di mitigare parzialmente le conseguenze di un simile, gravoso rincaro.

ma anche perché tradizionalmente vede una ripresa delle attività economiche proprio in vista delle spese natalizie: è un momento che gli imprenditori e le imprese aspettano per tutto l'anno, perché è evidente che la spesa delle famiglie aumenta notevolmente. Tuttavia, con questo provvedimento, si spera che non venga sacrificata ulteriormente la ripresa di molti settori economici, che proprio nel periodo natalizio riescono a dare sollievo alle loro casse, soprattutto dopo gli ultimi due anni complessivi, nei quali evidentemente c'è stato un calo notevolissimo. Il provvedimento del quale discutiamo oggi prevede uno stanziamento di fondi straordinari per arginare in qualche modo questi rincari, limitando soprattutto i costi fissi, rappresentati dagli oneri di sistema e dall'IVA. comprende l'azzeramento dei costi fissi per le piccole imprese e misure per le famiglie con i redditi più bassi, per non far pesare in alcun modo su queste categorie gli aumenti delle spese di consumo energetico, quindi avrà un effetto molto positivo sul Paese e sulla sua economia. Il provvedimento interviene a tutela di oltre 3 milioni di persone che già beneficiano del *bonus* energia.

reddito o di pensione di cittadinanza e utenti che si trovano in gravi condizioni di salute. Queste sono le categorie più fragili per le quali sono tendenzialmente azzerati gli effetti degli aumenti delle bollette.

Quanto al gas, per circa 2,5 milioni di persone che beneficiano del *bonus* sociale gas sono tendenzialmente azzerati gli effetti dell'aumento della bolletta.

effetti molto pesanti sull'economia delle famiglie. È però anche evidente la necessità di individuare nuovi interventi strutturali e di più ampio respiro, capaci davvero di fornire degli strumenti idonei

Gruppo Italia Viva-P.S.I., pertanto aderisce con entusiasmo a questo nuovo provvedimento del Governo che continua a prestare attenzione alle categorie più fragili.

del Parlamento a sostegno del Governo in questa direzione, con la consapevolezza che ci si sta muovendo nel verso giusto. L'Italia può riprendersi e ripartire in maniera adeguata se noi saremo capaci di svolgere quest'azione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione gli interventi di alcuni colleghi e non riesco a capire la visione

Lo sapete che questo aumento impatterà in maniera così grave che forse molte aziende dovranno chiudere, perché non potranno sostenere un aumento di costi così impattante? Chiedo dunque al Governo dei migliori: anziché finanziare con ulteriori risorse il reddito di cittadinanza, per far stare i nostri giovani a casa sul divano, magari a giocare alla *playstation*, perché non vi occupate delle politiche per il lavoro e del mantenimento del lavoro? Vi rendete conto che questo caro bollette impatterà in maniera enorme? Non vi viene una domanda spontanea e di buon senso? Capisco che ormai il buonsenso è molto lontano da questo Governo. Tutti voi, colleghi della maggioranza, vi riempite la bocca dell'aumento del PIL del 6 per cento per il prossimo anno,

Di tutto questo, però, non siete assolutamente preoccupati. Quindi, non riuscite a capire come questi miliardi di euro di aumento impatteranno in maniera devastante.

Questo dimostra che gli aumenti saranno ancora maggiori di quelli che prevediamo oggi. Ma - come ho già ricordato prima - le vostre scelte sono altre.

Questi sono problemi che, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, abbiamo sempre avuto ben presenti. È sempre quella stessa Europa che lascia da soli che, quando ci sarebbe bisogno di lei, non c'è, se non nei titoli e nelle dichiarazioni. È quell'Europa che pensa che Lampedusa sia il confine dell'Italia e non dell'Europa. È quell'Europa che si comporta nella stessa maniera con i migranti, pensando che il problema sia italiano e non europeo. Allora io credo veramente che dovreste fare un ragionamento più ampio. Bisognerebbe che voi capiste che c'è bisogno, c'è la necessità e l'urgenza di una riforma della politica energetica della nostra Nazione,

Noi di Fratelli d'Italia non vogliamo essere delle Cassandre. Noi di Fratelli d'Italia siamo dei patrioti e crediamo nella nostra Nazione. Ma mi dovete spiegare come fa questo Governo, un Governo degli opposti opposti che tiene insieme coloro che si erano contrapposti, a trovare delle soluzioni. No, colleghi: voi trovate delle mediazioni che non mettono mai al centro le risposte e le soluzioni per gli italiani. È per questo che annuncio il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia.

l'abbattimento del costo delle bollette, attraverso lo spostamento di alcune voci che sono al loro interno (gli oneri generali di sistema) e l'abbassamento delle aliquote IVA. Mi sembra chiaro, anche dalla discussione di oggi, che può apparire abbastanza inadeguato parlare di bollette di fronte all'importanza del dibattito sui temi energetici. C'è una discussione che interessa l'intero pianeta e che è stata affrontata poche settimane fa nel G20; è in corso ora la COP26 a Glasgow,

vede in qualche modo defilati alcuni soggetti decisivi per la definizione di azioni incisive per il futuro, e parlo di grandi Paesi come la Cina o l'India.

la questione energetica e del caro energia è stato uno dei temi affrontati in modo più preciso e adeguato dal punto di vista del nostro Paese,

e, quindi, rappresenta una difficoltà che pone ciascun Paese di fronte alle proprie capacità di affrontare il problema nella propria autonomia. Credo che questo sia un aspetto da sottolineare. Colleghi, la pandemia ci ha fatto fare - a livello europeo - un salto importante: abbiamo capito che c'è un'interdipendenza tra i Paesi nell'affrontare temi sovranazionali,

che la pandemia ci ha fatto capire che i vaccini sono la risposta che andava presa, affrontata e portata avanti in modo comunitario, sul tema dell'energia e della transizione ecologica questa consapevolezza ancora non l'abbiamo, e capiamo che dobbiamo fare passi importanti. Su questo voglio sottolineare un aspetto che deve essere una nostra consapevolezza: la transizione ecologica non è la transizione energetica *tout court*; è la transizione del nostro sistema produttivo. Questo è il tema che dovremmo affrontare. Riconosco al MoVimento 5 Stelle di aver portato sensibilità rispetto ai temi dell'ecologia, della transizione ecologica e del rispetto del pianeta, con forza all'interno dell'istituzione; una forza che fino a quel momento non c'era ancora stata. Dopodiché, dobbiamo costruire questa transizione; abbiamo il compito di tracciare il percorso che arrivi all'obiettivo, che è la decarbonizzazione. Quell'obiettivo è da raggiungere per esserci in un pianeta vivo, ma dobbiamo arrivarci con un sistema produttivo e sociale vivo. Allora, questo deve essere il percorso che dobbiamo tracciare. pochi giorni fa il capo della Volkswagen ha annunciato che ci saranno 30000 licenziamenti su 100.000 dipendenti totali nel settore automobilistico in Germania. È un annuncio che vale oggi per il prossimo anno. Costruire il percorso che dà una sostenibilità integrale alla transizione energetica significa tenere conto del complesso delle azioni che bisogna porre in essere per dare alla transizione ecologica il percorso giusto. La transizione non è un salto; il salto non è sostenibile. La transizione è il percorso che dobbiamo costruire.

la transizione va finanziata e sostenuta negli investimenti che devono essere fatti sia per incentivare le nuove tecnologie sia per sostenere gli investimenti di trasformazione del sistema produttivo. Sul punto dobbiamo arrivare a delle sintesi che troviamo la dimensione della transizione nella capacità di individuare le varie fonti che ci devono accompagnare e devono consentirci di rendere sostenibile la transizione ecologica ed energetica. È chiaro allora che non possiamo immaginarci di arrivare al 2050

ad avere competitività attraverso le fonti tradizionali mentre le andiamo a sostituire, attraverso un percorso di investimento e anche di avanzamento tecnologico, con le fonti che non danno impatto

dovrebbe assorbire il 40 per cento delle risorse mondiali del gas presenti nel pianeta. Abbiamo necessità di portare al tavolo della discussione soggetti importanti come la Cina perché, diversamente, tutti i nostri sforzi saranno non solo inutili, ma mineranno la nostra capacità di rimanere sul mercato con il sistema produttivo.

all'incremento dei costi, che in parte è congiunturale e, in parte, strutturale. Credo però che non dobbiamo perdere l'occasione di iniziare in modo significativo con il Governo una riflessione che ci faccia costruire il percorso

sacrosanto; è uno di quei rari casi in cui evidentemente i criteri di urgenza e necessità trovano forma concreta in un intervento normativo di iniziativa governativa. La riduzione del costo delle bollette in relazione all'ultimo trimestre dell'anno in corso è stato, un intervento necessitato dalle notorie dinamiche dei prezzi delle bollette, soprattutto di elettricità e gas, dovute agli eventi - notori anch'essi - di ambito geopolitico e dei mercati internazionali dell'energia. Se le previsioni di aumento in relazione al trimestre in questione prevedevano un aumento dell'energia elettrica del 45 per cento e quello del gas del 30 per cento, grazie a questo intervento

cui possiamo far riferimento per dire che la politica c'è, nella misura in cui è possibile farlo. L'intervento del Governo e quello nostro parlamentare sono un atto di testimonianza e di vicinanza al tessuto imprenditoriale e alle famiglie italiane. L'abbattimento degli oneri di sistema - su cui mi soffermerò - avviene peraltro mediante una parte dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO₂. Sappiamo che, per quanto riguarda l'elettricità, saranno annullati sostanzialmente gli oneri di sistema per il trimestre in questione, fino a una potenza massima di 16,5

l'onere fiscale dell'IVA al 5 per cento, con i risparmi conseguenti. Ancor più apprezzabile è l'intervento previsto nell'articolo 3, dove il Governo e il Parlamento si preoccupano, dei *bonus* sociali, di azzerare gli aumenti per le categorie economicamente svantaggiate e i clienti domestici in gravi condizioni di salute. Si tratta quindi di un intervento i presupposti di necessità e urgenza; il contenuto è condivisibile. Venendo a qualche riferimento più generale, in base anche al dibattito che si è svolto finora sia in fase di discussione generale che di dichiarazioni di voto, sembriamo essere tutti concordi nel dire che la via d'uscita, al di là di provvedimenti emergenziali seppur necessitati come questo, è pensare a riforme strutturali che incidano nel più breve tempo possibile (il che non vuol dire domani, perché magari il giorno dopo non è possibile). Gli interventi strutturali che la politica energetica nazionale deve deve perseguire sono quelli dell'abbandono delle fonti fossili: ce lo stiamo dicendo tutti, ma poi nel concreto dobbiamo capire quanto e come siamo disposti a scommettere e a credere veramente che il potenziamento delle fonti di energia rinnovabile, pur con i propri limiti e difetti, sia l'unica via che ci consentirà di staccare il cordone ombelicale che lega il nostro Paese,

I colleghi dell'opposizione di Fratelli d'Italia hanno evocato un piano nazionale dell'energia, ma questo c'è e si sta costruendo giorno dopo giorno, grazie anche alla grande opportunità del PNRR. Dobbiamo aumentare grandemente la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, quello intelligente, quello fatto sui tetti, quello che utilizza le nuove tecnologie dell'agrovoltaico compatibili con la produzione agricola. Dobbiamo aumentare la produzione idroelettrica con l'eolico, soprattutto *offshore*, poco o per nulla impattante a livello visivo. Dobbiamo rafforzare con grande velocità, semplificando il semplificabile - come in parte è stato già fatto - questo tipo di direzione. La tematica dell'accumulo viene in risalto, come giustamente ricordava in discussione si stima che ci siano duecento bacini idrografici che possono essere potenziati per costruire e ottimizzare sistemi di accumulo per l'idroelettrico. A me piace ricordare anche in questa occasione che si sta sviluppando un'altra tecnologia e che grandi investimenti si stanno spostando verso il cosiddetto idrogeno verde, cioè quello prodotto da fonti rinnovabili, che può essere il vettore energetico che aiuterà la risoluzione dei problemi dell'accumulo di energia elettrica che - come sappiamo - deve avere un consumo immediato e, per essere conservata, necessita di sistemi a batteria molto costosi; l'idroelettrico ha limiti fisici. È curioso vedere che si stanno sperimentando anche altri sistemi di accumulo energetico, come il cosiddetto volt gravitazionale: enormi gru sollevano, portando in basso e in alto grandi blocchi di cemento di 35 tonnellate, utilizzando il movimento degli argani per produrre energia elettrica rinnovabile in sovrapproduzione per sollevare i pesi e poi, lasciandoli cadere, producono a loro volta energia che attiva turbine e si produce energia elettrica. Questo però lasciamolo a chi lo sta sperimentando e sta investendo in Paesi

2019 ha già redatto alcune soluzioni che potrebbero portarci notevoli risparmi di spesa, da investire per l'ottimizzazione ecologica ed energetica del Paese, intervenendo su circa 34,6 miliardi non da da un giorno all'altro e tutti insieme, ma in maniera intelligente, iniziando a eliminare i sussidi che diamo ancora per trivellazioni o fondi di ricerca per il gas, il carbone e il petrolio.

si potrebbe togliere, e cioè l'incentivo per le caldaie a gas. Pur essendo quelle di ultima generazione più performanti rispetto alle vecchie caldaie a gas, consumano ancora gas, e cioè ci tengono ancora attaccati alle fonti energetiche fossili, che ci vedono costretti a essere ancora dipendenti dall'approvvigionamento straniero e anche non ecologico, per le notorie perdite che il sistema del gas comporta.

Forza Italia voterà a favore del provvedimento in discussione, apprezzando lo sforzo che il Governo ha sostenuto in tempi anche molto rapidi per sterilizzare l'aumento del conto energia. Tuttavia, non possiamo assolutamente non evidenziare una seria preoccupazione con riferimento ad alcuni dati che, se si dovessero verificare secondo le previsioni, avrebbero ripercussioni fortemente negative sulle famiglie più povere, ma anche su quelle che hanno avuto serie difficoltà negli ultimi due anni, attingendo in parte significativa ai loro risparmi per poter andare avanti, così come sulla piccola e media impresa. Io credo che, per onestà intellettuale e soprattutto per avviare una riflessione molto pacata su questi argomenti, sia doveroso ricordare alcune cifre. cifre. Se dovessero rimanere invariate le aliquote tariffarie, il costo del gas naturale nel corso del 2022 sarebbe di circa 9,5 miliardi. Questo perché le quotazioni del gas sono doppie

rispetto a quelle del periodo pre-Covid, anche se la Russia - per essere molto chiari - ha riaperto i rubinetti. Per la verità ci stiamo - per così dire - un po' strappando tali forniture tra Cina e Europa. Ricordo che la Cina - collega Buccarella - non è un continente, ma - grazie a Dio - ancora solo una Nazione, per quanto molto grande.

al fatto che esiste una forbice tra offerta e domanda di 4-5 punti percentuali. Risponde anche al fatto che sta attingendo alle riserve. Durante il periodo del Covid-19 non ci sono stati investimenti e questo è un altro elemento da attenzionare.

in equilibrio. L'energia all'Italia costa 4-5 volte di più di quello che costa agli Stati Uniti. La nostra industria è estremamente energivora e produciamo molta CO2, dovendo pagare anche le giuste tasse per le

oramai da tantissimi anni. Purtroppo le cose non si improvvisano dalla sera alla mattina: ci vuole tempo per approntare gli investimenti, per dare una risposta strutturale in termini di *mix* energetico,

il danno da mancati ricavi e da costi di ricostruzione dovuti a eventi atmosferici estremi potrebbe essere nell'ordine di un paio di miliardi. Dico questo perché tutte le infrastrutture

si ripercuoteranno necessariamente sul prezzo finale che dovrà pagare l'utente.

Così come non si può essere ancora in ritardo su una dipendenza energetica che il nostro Paese ha dall'estero. È esattamente la stessa dipendenza energetica che ha anche l'Europa, correttamente il collega di Fratelli d'Italia. Ursula von der Leyen ha detto che il 90 per cento del gas naturale consumato in Europa viene importato e questo non è più sostenibile. Bisogna assolutamente pianificare in termini strategici gli approvvigionamenti e l'autosufficienza. *(Applausi)*. Chiaramente tutto questo va di pari passo con una revisione del metodo

dentro la fiscalità generale. E allora, con un atto di grande coraggio, secondo me, il nostro Governo, guidato dal nostro autorevole *Premier*, dovrebbe avviare, anche a livello di Commissione europea, il confronto sulla tariffa unica.

un'altra piccola riflessione, collegandomi al prossimo disegno di legge di bilancio, sulla crescita economica. Sappiamo che la crescita economica è seriamente compromessa e questo va detto.

tamponare gli aumenti dei prezzi, non riusciremo a sostenere la domanda interna, perché necessariamente, con meno soldi, i consumi domestici deflettono. Un'ultima considerazione, dopo che il relatore ha fortemente espresso le sue critiche sul nucleare. Questa mia considerazione si rivolge al sistema universitario. Qualche giorno fa abbiamo sentito il coordinatore di tutti i rettori, il professor Resta, esortare a considerare l'università come un'organizzazione a fianco dello Stato e dei privati, in un momento estremamente complicato, in cui stiamo attraversando

con una grande opera di formazione dei futuri ingegneri, dei futuri biologi e dei futuri scienziati, ci aiuti a capire (perché la politica deve solo capire e poi deve assumersi la responsabilità delle scelte)

in pochi mesi è la seconda volta che il Governo interviene per mitigare il caro energia. A maggio l'aumento del 30 per cento dei prezzi del gas legato alla ripresa delle economie e l'aumento dei prezzi di emissioni della CO2 per effetto della decarbonizzazione imposta dalla UE hanno portato il Governo a stanziare 1,2 miliardi per contenere per il terzo trimestre l'incremento al 9,9 per cento della bolletta della luce, che diversamente sarebbe stato del 20 Le quotazioni, però, della CO2 e soprattutto del gas hanno continuato impetuosamente a crescere e da settembre si sono impennate. Dalla burrasca ci siamo trovati nella tempesta perfetta: il gas nell'ultimo anno è a più 400 per cento e ha spinto i prezzi elettrici a livello *record*. Il Governo, intervenendo con questo decreto, stanziando 3,5 miliardi, ha consentito in questo quarto trimestre di ridurre l'impatto del 30 per cento per l'elettricità e del 14,4 per cento per il gas. In assenza della misura, gli aumenti sarebbero stati rispettivamente del 45 per cento e del 30 per cento. Si sono ridotti gli oneri in bolletta e l'IVA per il gas a 35 milioni di clienti domestici, microimprese e piccole imprese

è stata un'operazione straordinaria, assolutamente necessaria, ma che purtroppo non ha evitato la batosta del caro bollette a molti. Penso, per esempio, agli utenti del teleriscaldamento e a quelli del gas naturale per autotrazione, per il quale non è stata riconosciuta l'IVA agevolata al 5 Oltre ai mezzi pesanti, stiamo parlando di un milione di auto a metano che oggi rispetto a un anno fa pagano il combustibile il 70 per cento in più. Sono in ginocchio loro e l'intera filiera. Sono in difficoltà i sindaci per i bilanci del proprio Comune e, in generale, tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli ospedali. Sono in difficoltà le medie e grandi imprese e quelle energivore del gas. Alcune imprese hanno aperto linee di credito con le banche per pagare le bollette. Penso all'accordo fatto da Confindustria Lecco-Sondrio. Altre imprese, nonostante siano pieni di ordini, stanno rallentando la produzione e talune si sono fermate perché produrre è diventato troppo costoso, come deciso da otto fornaci del distretto del vetro di Murano. Insomma, sono a rischio tanti posti di lavoro e ci saranno problemi sociali. A queste realtà in crisi la Lega ha cercato di dare risposte con emendamenti, ma il Governo, rinnovando l'impegno di intervenire anche con la manovra, in fase di conversione del decreto non ha previsto risorse aggiuntive e tutti gli emendamenti onerosi sono stati purtroppo respinti. Noi, però, li ripresenteremo in manovra. Il fenomeno del caro energia non è ovviamente solo italiano; ha dimensione internazionale, ma l'Italia soffre molto di più perché paga inefficienze mai risolte e scelte discutibili fatte in passato come il conto energia che ha sostenuto gli impianti rinnovabili, dove sono state aumentate le speculazioni, sono aumentati gli oneri di sistema e non si è creata una filiera nel nostro Paese. I pesanti aumenti indeboliscono la competitività delle nostre imprese e colpiscono le famiglie, magari non tutte direttamente in bolletta grazie all'intervento governativo, ma indirettamente per per l'inevitabile aumenti dei prezzi dei beni di consumo legati agli aumenti dei costi di produzione. I rischi che venga frenata la ripartenza *post* pandemia e che parta l'inflazione sono altissimi. La situazione è sempre più grave, sempre meno congiunturale e rischia di essere strutturale. Cerco di mostrarvelo. (*Il senatore Arrigoni sono riportati i prezzi medi giornalieri dell'energia elettrica in Europa nel mese di settembre: più scuro è il colore, più alto è il prezzo dell'energia. Faccio due rilievi: l'Italia ha il triste primato del prezzo più alto. Noi, infatti, eravamo a 159 euro a megawattora, la Francia a 135 (meno 15 per cento) e la Germania a 128 (meno 20 Segnalo che nel 2019 il prezzo era da noi 52 euro, cioè un terzo. Evidenzio che proprio con i prezzi di settembre il Governo ha stanziato 3,5 miliardi per ridurre gli aumenti in bolletta. In questo secondo grafico, notate invece i prezzi del mese scorso, ottobre: i colori sono più scuri e questo deve far preoccupare. Faccio alcuni rilievi. L'Italia mantiene il triste primato del prezzo di energia elettrica più alto. Rispetto alla media di settembre, quando il prezzo italiano era di 159 euro a megawattora, quello medio di ottobre è salito a 218 (l'aumento è del 37

Forse perché la Germania - ma la mia è una domanda retorica - ha un ampio *mix* energetico con nucleare al 13 per cento, carbone e lignite al 35 Peraltro, noi abbiamo deciso di spegnere le centrali a carbone entro il 2025, la Germania forse al 2038. Hanno tante biomasse che noi invece non sviluppiamo e poi hanno il gas, che ricevono direttamente dalla Russia, con il Nord Stream, che fra poco raddoppierà.

ha rilanciato la costruzione di reattori nucleari ad impatto zero. Appare evidente che stanno meglio i Paesi che non hanno ancora rinunciato al carbone e che sfruttano il nucleare, peraltro evitando l'emissione di milioni e milioni di tonnellate di CO2 al mondo. Quali conclusioni traiamo? Che la competitività delle nostre imprese e i bilanci delle famiglie italiane si stanno sempre più compromettendo e che i 2 miliardi stanziati in legge di bilancio per limitare il caro bollette nel primo trimestre 2022 sono decisamente insufficienti e lontani dall'avere effetto di mitigazione pari a questo trimestre. Poiché l'inverno si sta avvicinando, è il caso di preoccuparsene. Le cause di questa drammatica situazione italiana sono anche da ricercare nel nostro particolare *mix* energetico e nell'eccessiva dipendenza energetica dall'estero: per il gas è del 95 per cento e ci permettiamo il lusso, ipocritamente, di non sfruttare il nostro gas a chilometro zero, più pulito e sfruttabile a emissioni ridotte rispetto a quello che per almeno trent'anni saremo costretti ad importare. Cosa fare, dunque? Nell'immediato - ripeto - serve un'iniezione molto maggiore di 2 miliardi e allargare la platea dei beneficiari e poi bisogna intervenire strutturalmente e ripensare alla politica energetica del Paese. L'Italia non può aspettare l'Europa che, dopo l'ubriacatura del solo rinnovabile e solo idrogeno verde, purtroppo è divisa su come affrontare il caro energia e forse solo a dicembre deciderà qualcosa. La nostra ricetta non può essere quella dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, che spingono solo su fotovoltaico ed eolico. A proposito, le comunità energetiche non sono solo affare vostro, abbiamo contribuito anche noi come Lega ad introdurle. Anche se i sistemi di accumulo saranno sviluppati tecnologicamente, non si risolve il problema della loro non programmabilità. Vedete, il problema di queste rinnovabili non si manifesta nei costi bassi di produzione dell'energia elettrica, ma nei costi altissimi della non produzione, non solo quando non c'è il sole o il vento, ma soprattutto in inverno e con le sole rinnovabili non si può rispondere alla domanda di energia crescente. Occorre dunque tornare ad investire con biomasse, geotermia e idroelettrico, deflusso ecologico permettendo. Occorre - ed è ormai indifferibile - abbattere strutturalmente gli oneri di sistema che pesano 15 miliardi e spostarli nella fiscalità generale. Occorre - è stato oggetto di diversi ordini del giorno della Lega approvati - incrementare l'efficacia del servizio di interrompibilità per le imprese energivore del gas, fondamentale con l'inverno alle porte e poi agire in sede comunitaria per definire un regolamento che stabilisca regole comuni per gestire in sicurezza gli approvvigionamenti del gas e gli stoccaggi e agire nel pacchetto sulla finanza sostenibile e sulla tassonomia per inserire il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica

Occorre infine assumersi la responsabilità, per sfruttare il nostro gas naturale e ridurre la nostra dipendenza energetica, di investire per diversificare le fonti di approvvigionamento decarbonizzare - sì - con nuovi alberi, caro collega Anastasi, ma anche con la cattura e lo stoccaggio della CO2 e non chiudersi allo sviluppo e alla ricerca del nucleare di quarta generazione. In sintesi, occorre abbandonare l'ambientalismo ideologico anti-impresa e procedere

senatore Arrigoni, sulla tassonomia noi ci siamo astenuti e le ricordo che sul nucleare ci sono stati ben due *referendum* in Italia. *(Applausi)*. Ad ogni modo, oggi parliamo di bollette. La pandemia continua a produrre effetti nefasti sulla nostra economia. Superata la fase acuta, siamo oggi chiamati anche a fronteggiare le ricadute della progressiva ripartenza economica, come lo straordinario aumento dei prezzi di energia elettrica e gas. Tra i fattori scatenanti che hanno contribuito all'acuirsi di questo fenomeno vi è sicuramente la tendenza di forte crescita delle quotazioni delle principali materie prime energetiche, arrivate ai massimi storici e ancora in forte aumento per la ripresa delle economie mondiali a seguito dei ribassi dovuti alla pandemia e alle difficoltà nelle filiere di approvvigionamento.

in aumento anche i prezzi correlati al costo dell'anidride carbonica, che ha raggiunto il *record* di quasi 60 euro a tonnellata. Tutto ciò si traduce in aumenti intollerabili in bolletta che, per una famiglia tipo, sono stati stimati in circa 145 euro all'anno per quella dell'elettricità e 155 euro per quella del gas.

a causa dell'offerta che continuerà a contrarsi. Se le ragioni degli aumenti sono da rinvenire nelle citate concause di natura squisitamente internazionale, le conseguenze sono invece tutte interne al nostro Paese, condizionano la nostra economia e si ripercuotono direttamente sui consumatori finali. Da un lato, ci sono le famiglie (specialmente quelle meno abbienti e del ceto medio), che rischiano di essere sempre più oppresse da una pressione fiscale non più sostenibile.

A ciò si aggiungono l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021 per circa 6 milioni di microimprese e circa 29 milioni di clienti domestici, nonché la riduzione dell'IVA per tutti gli utenti del gas naturale. Come già detto, si tratta di un primo passo certamente indefettibile, ma al tempo stesso provvisorio e pertanto anche non del tutto sufficiente. Quello di oggi, quindi, non può che essere un primo provvedimento che dovrà condurre verso un sentiero lastricato di azioni sinergiche da parte di tutti i Dicasteri interessati, partendo dalle necessarie iniziative volte a contenere alla radice il fenomeno dei rincari a livello internazionale e, parallelamente, con interventi economici mirati e concreti diretti al ceto medio e alle imprese di maggiori dimensioni. Mi riferisco in particolare alle medie e grandi imprese energivore, come quelle del settore ceramico, le cartiere o le fonderie, che a causa degli aumenti vedono lievitare i costi della propria produzione di diversi milioni di euro al mese e rischiano conseguenze potenzialmente devastanti, in alcuni casi addirittura la chiusura. Dobbiamo intervenire senza indugio, dando buone prospettive, affinché gli occupati abbiano una stabilità e siano in grado di sostenere le proprie famiglie e affinché gli imprenditori continuino ad innovare e ricercare per restare all'avanguardia: il *made in Italy* si difende anche così. Ritengo quindi necessario che vengano realizzate iniziative urgenti, anche in considerazione del fatto che gli interventi calmierati già adottati si esauriranno molto presto, esattamente al termine del quarto trimestre dell'anno. Sin dalla scorsa estate, il MoVimento 5 Stelle è stata la prima forza politica a chiedere un intervento immediato contro il caro bollette. Lo abbiamo fatto in via ufficiale con una mozione di maggioranza, a prima firma del capogruppo alla Camera dei elencando anche i possibili interventi per affrontare strutturalmente il fenomeno. Siamo stati noi i primi a batterci anche per abbassare, in via generale, i costi elevati delle bollette. Da un lato continuiamo a sostenere la necessità di intervenire urgentemente sugli oneri di sistema, ma occorre tracciare anche un altro sentiero, che porti alla vera tradizione ecologica. un cammino che abbiamo già intrapreso, adottando misure concrete, come il superbonus 110 per cento e le comunità energetiche, in grado di ridurre immediatamente i consumi e quindi anche le emissioni a tutela dell'ambiente e di generare un risparmio immediato per i cittadini. Gli investimenti sulle rinnovabili, sull'efficientamento energetico, sulla diffusione e sui sistemi di accumulo sono obiettivi non più rinviabili, per i quali dovremo batterci fianco a fianco, tutti insieme. L'alternativa è quella di continuare a dipendere dalle fonti fossili e quindi soggiacere proprio a quel ricatto economico che oggi rischia di mettere in ginocchio milioni di cittadini e migliaia di imprese e che ci costringe a stanziare urgentemente ingenti risorse, che di certo non generano un ritorno economico positivo per la nostra economia.

Ma c'è un «ma»: dalle ultime notizie, sembra infatti che il Governo non sia intenzionato a dare seguito agli impegni presi in quest'Aula su una proroga generalizzata fino al 2023. 2023. Vorrei dire a tutti i colleghi che non possiamo lamentarci del fatto che il Parlamento venga puntualmente esautorato, quando addirittura, pur essendo tutti concordi su un tema non divisivo, non riusciamo a convincere il Governo a seguire l'indirizzo politico espresso dal Parlamento. Le premesse non sono affatto rassicuranti: su una manovra di bilancio di 30 miliardi di euro, non si può lasciare un margine di intervento così stretto al Parlamento, compromettendone, sebbene parzialmente, le prerogative. In particolare per le modifiche economicamente più rilevanti non c'è margine: o andiamo tutti ad annusare i meloni, riconoscendo la nostra irrilevanza, o siamo conseguenti e teniamo il punto nelle Commissioni. *(Applausi)*. Il Parlamento vuole il superbouns: punto! Invece accade che si tenti di bloccarne la lievitazione, disorientando cittadini ed imprese, che rinunciano dopo aver investito tempo e denari nelle progettazioni. Se lo vogliamo tutti, il risultato si porta a casa. Mi pare di essere stato chiaro: si agisca nelle Commissioni o si taccia per sempre! Chiedo pertanto che sia il Governo a trovare le dovute coperture, per assicurare la proroga del superbonus, almeno fino al 2023, eliminando soglie ISEE e tutte le formule e le eccezioni che rischiano soltanto di creare incertezze e difficoltà applicative. Con queste premesse e con l'auspicio che questo sia soltanto il primo dei provvedimenti che si renderanno necessari per salvaguardare cittadini e imprese, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

Signor Presidente, non possiamo non vedere gli sforzi del Governo nel fare il minimo del minimo, di fronte a un rincaro spaventoso e insostenibile per imprese e famiglie. Sotto la soglia prevista da questo intervento era impossibile andare; però tutto si ferma qui. Per questo ci asterremo. Dopo questo *pit stop* non c'è alcunché di strutturale che consenta alle piccole e medie imprese e alle famiglie di pagare bollette del gas e della luce meno care. Ve lo dico soprattutto alla luce delle intenzioni di switchare verso l'elettrico e verso le fonti rinnovabili, tant'è che, alla luce di quel che fate (o meglio di quello che non fate), ritengo che le rivoluzioni verdi saranno soltanto per chi ha portafogli ricchi e per chi ha bilanci floridi. Ho l'impressione che, fintanto che i grossi gruppi non vi consegneranno le norme da approvare (perché ve le hanno scritte loro) e gli interventi da apportare (che vanno bene a loro), voi starete in *stand-by*. Vi avevamo proposto di premiare in via definitiva, con bollette meno care, coloro che già consumano energia da fonti rinnovabili. Invece voi cosa fate? la proposta, perché ci contestate il fatto che non è una misura a termine. In poche parole abbiamo sbagliato, secondo voi, a volere una norma che premiasse una volta per tutte chi consuma responsabilmente energia pulita. Tralascio anche il vostro voto contrario di fronte alla nostra proposta di rimborsare le bollette di chi ha avuto attività imprenditoriali chiuse durante il *lockdown* e di metterle in carico alle grandi società di distribuzione, che proprio nel periodo del *lockdown* hanno aumentato i loro profitti. Quindi, ricapitolando, la morale della vostra politica è: incentivi e premi per gli energivori (per i grandi) e bollette sempre care per famiglie e PMI. Quello che avete fatto - ripeto - è solo il minimo sostegno possibile.

l'auspicio è che vediamo risultati concreti del lavoro che dovrebbe essere fatto dalla stessa e che effettivamente ci si inizi a muovere in maniera un po' più concreta, in modo tale che i risultati vengano portati che i risultati vengano portati anche all'esame di quest'Assemblea. Com'è noto, c'è stata una discussione sulla data di termine della proroga,

che risulta essere una delle pagine più buie del nostro Paese, tanto che, se raccontassimo i fatti a chi non ne conoscesse minimamente l'esistenza, penserebbe a un film dell'orrore o comunque a una vicenda che non potrebbe accadere nel nostro Paese, tanto meno nella nostra civilissima Toscana. È vero che stiamo discutendo di una proroga, sottolineo necessaria, ma credo sia opportuno ricordare a noi tutti i punti fondamentali di questa vicenda. Il luogo, Vicchio di Mugello, una vallata dell'Appennino toscano, in provincia di Firenze: un luogo dove per circa trent'anni sono stati accolti minori in affidamento, allontanati da famiglie con gravi problemi; un luogo dove sono stati commessi gravi abusi sessuali e violenze su minori; un luogo dove si predicava o si attuava una teoria educativa, sociale, un modello di famiglia - sinceramente non saprei come definirlo - voluto e gestito da un certo Fiesoli, capo di quella comunità. Cito le stesse parole che ho usato in quest'Aula quando votammo la legge istitutiva della Commissione: "Il Forteto" è stata una setta totalizzante in cui si è annullata la personalità dei soggetti, di ragazzi con gravi problemi, e si sono rovinate decine, centinaia di famiglie e di persone, perché al "Forteto" non ci sono stati soltanto gravissimi abusi su minori, le violenze, le botte, i rapporti sessuali completi messi in atto dal Fiesoli; in quel luogo c'erano bambini che venivano fatti alzare all'alba per andare a lavorare, prima di essere portati a scuola, per fare un formaggio che magari mangiavano i tanti ospiti illustri - da politici a magistrati - che hanno frequentato la struttura. Dopo le due Commissioni di inchiesta della Regione Toscana e i processi, che hanno visto condanne, è emerso che in quel luogo è stato permesso di tutto nel silenzio e con la connivenza della politica, della magistratura, dei vertici socio-sanitari; con l'avallo e l'aiuto della Regione Toscana e delle amministrazioni locali, che per anni hanno considerato "Il Forteto" un esempio, finanziandolo e promuovendolo. *(Applausi).* Ancora oggi le responsabilità politiche non sono definite, non è ancora ben definito quale sia stato il meccanismo che ha creato il corto circuito del sistema; uno scaricabarile delle responsabilità fra chi doveva controllare e aveva il dovere di tutelare e proteggere quelle che allora sono state giovani vittime. vittime. In questi mesi abbiamo ascoltato molti di quegli attori: le vittime, i consulenti. Ancora oggi ci chiediamo come è possibile che sia successo tutto ciò, chi ha protetto Fiesoli. È possibile che i magistrati, i politici, gli operatori che hanno avuto a che fare con "Il Forteto" abbiano agito tutti in buona fede? È possibile che nessuno si sia mai accorto di nulla? Ancora queste domande non hanno una risposta completa e compiuta. Dobbiamo andare a fondo di questa vicenda, e per questo occorre altro tempo; troppi sono ancora gli angoli bui. Soprattutto mi rivolgo al Presidente della Commissione e ai colleghi: usiamo bene il tempo che ci viene nuovamente concesso per andare nel vivo della questione.

rappresenta la parte più estrema e drammatica delle vicende degli affidamenti - purtroppo non unica nella sua drammaticità, penso ad esempio alla vicenda di Bibbiano - occorre ricordare quanto sia necessario approfondire in misura ancora maggiore il tema generale e delicato degli affidi. Per questi motivi e molti altri annuncio il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia.

È una Commissione che chiede responsabilità; noi siamo qui per questo, l'abbiamo sempre votata e abbiamo partecipato in tal senso. Dispiace che il senatore La Pietra abbia svolto già una relazione

si arrivi a votare una relazione su questo fatto increscioso, drammatico e tragico che riguarda sicuramente tutta l'Italia, ma in particolare una zona della Toscana, che mi è particolarmente cara. Si arrivi, per per il rispetto che è dovuto a tutti gli interessati, a tutte le vittime dirette e indirette, a votare una relazione il prima possibile,

qualcosa di non chiaro. La Commissione sta lavorando, ma non è tollerabile che ci sia ancora, in questo momento in cui, lo ricordo, votiamo solo la proroga, la strumentalizzazione di chi pensa di avere in Assemblea già una relazione sul tema. che ci chiama, senatore La Pietra, ad avere responsabilità verso le vittime. Votiamo intanto la proroga e poi diremo nella relazione tutto quello che abbiamo riscontrato, ognuno nelle sue posizioni.

i senatori presenti hanno deciso di assumere per continuare a cercare quella verità che per troppo tempo, per decenni, è stata nascosta. In questi mesi, nonostante l'attività della Commissione abbia subito rallentamenti, abbiamo avuto modo di appurare che gli appelli lanciati negli anni non erano stati vani. Ricordo che il giudice Bouchard dopo decenni di impunità ha presieduto il collegio che ha condannato Fiesoli, peraltro già inquisito nel 1978 per pedofilia,

che stabiliva tutta una serie di caratteristiche per aprire una comunità. Il problema è che qualunque fosse l'accezione che si volesse dare all'esperienza del Forteto nell'accoglienza del minore, mancavano totalmente i requisiti*.* Nessun tipo di autorizzazione, di procedura e di verifica è mai stata fatta sulle caratteristiche di quella struttura». Se le pratiche fossero state fatte, quella cooperativa non sarebbe durata neanche un giorno. *(Applausi)*. Queste le parole del giudice. Non c'era però interesse ad approfondire cosa accadeva perché i minori avevano sia condizioni difficili per una collocazione diversa sia perché il Forteto non chiedeva rette e per le Istituzioni rappresentava una soluzione davvero conveniente. Non chiedeva rette, ma aveva finanziamenti per milioni di euro all'anno. Ricordo ancora quando, nella XVI legislatura, Rodolfo Fiesoli venne in Senato a presentare il suo libro, presentato da una forza politica. Un vero e proprio *j'accuse* nei confronti del sistema che ha causato *blackout* e ha provocato danni a decine e decine di vittime minori, e non solo. Il caso di cui ci stiamo occupando ha bisogno di tempo e spazio per il dibattito, affinché lo Stato possa recuperare il rispetto che negli anni ha perso nel silenzio e nell'omertà. Sull'uscio di questa comunità si sono fermate, senza entrare, le istituzioni, i controlli dei servizi sociali, la magistratura, i giornalisti, accontentandosi della versione che dall'interno veniva fornita. Una sorta di zona franca da cui lo Stato ha deciso di distogliere lo sguardo, di far finta che questa comunità, queste persone e quanto avveniva in quel luogo non esistessero. Di ottanta bambini, quattordici si sono suicidati. approfondire, prima per coscienza individuale, poi per tutti coloro che rappresentiamo, gli italiani. Per queste ragioni, mi auguro che la Commissione possa recuperare il tempo perduto a causa dell'emergenza sanitaria, preparandosi anche a una vera riforma normativa che riguardi le case famiglia. In tutta Italia ci sono casi, forse non della gravità del Forteto, che chiedono vendetta e, soprattutto, controlli. Forza Italia vuole chiarezza per le famiglie e i bambini che soffrono tremendamente perché lontani dalla loro quotidianità. Questo per non parlare del giro di soldi di soldi denunciato, che passa tra alcuni assistenti sociali, giudici minorili e case famiglia, com'è emerso nella Commissione infanzia nella scorsa legislatura.

A lei va il mio pensiero, cara collega. Ricordiamo allora il fatto: una comunità agricola fondata nel 1977, che poi dal 1978

la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia perché ha dato ancora dei bambini a quella comunità agricola; Finalmente nel 2015 vi siete arresi, perché è stata finalmente chiusa. Leggo alcune delle motivazioni della sentenza, perché è giusto ricordarle in quest'Aula; bisognerebbe fare un film su questa vicenda. sentenza del tribunale: «nel condizionare le scelte di voto» - quello facevano - «in occasione di elezioni politiche ed amministrative»;

il non affetto tra genitori e figli. Questo è successo. La scarcerazione dei due condannati veniva festeggiata con politici e sindacati. Forse voi avete paura dei nomi di questi! Vengo alle conclusioni perché la sentenza è pubblica e poi ne vedremo veramente delle belle. Ieri, come ha detto una mia collega, il presidente della sezione penale del tribunale di Torino ha ricordato una cosa che vorrei

delle domande su come sia potuto accadere questo. Concludo ricordando che la Commissione ha accumulato 70.000 pagine. Abbiamo fatto tantissime audizioni. Vorrei ringraziare di cuore il comandante della Guardia di finanza

alle istituzioni rispetto a tutto quello che abbiamo ascoltato, nelle tantissime audizioni svolte, da parte delle vittime, degli assistenti sociali e dei magistrati, perché non si può sentire una persona dire che i bambini dovevano essere mandati da qualche parte o assegnati a qualcuno: è questo il problema. La proroga non c'entra nulla con il fatto di fare qualcosa sul sistema degli affidi, perché in questa legislatura abbiamo istituito anche una Commissione apposita per il sistema degli affidi, che deve collaborare con noi; possiamo partire subito, appena conclusa la sessione di bilancio. Mettiamoci al lavoro sulla questione degli affidi, ma non togliamo la possibilità, mettendo fretta, di capire realmente cosa è successo al «Forteto» e dare le colpe a chi le ha, senza fare di tutta l'erba un fascio. Il MoVimento 5 Stelle dal 2013 in quest'Aula ha sempre portato avanti l'idea di tutelare le vittime e cercare di indagare il più possibile. Quindi, il nostro voto sarà favorevole al

Signor Presidente, ho chiesto la parola per ricordare una figura, una senatrice: cent'anni fa, l'11 novembre del 1921, nasceva Alessandra Codazzi, partigiana, sindacalista della CISL e poi senatrice della Democrazia Cristiana nell'VIII, IX e X legislatura. Ho avuto l'onore di conoscere Sandra, che andavo a trovare nella sua abitazione nel quartiere Africano di Roma. Davanti a un buon tè, servito dalla sua figura minuta ma forte di animo e di spirito, mi dispensava con immensa generosità e competenza consigli per la mia attività di allora, responsabile del Coordinamento Mi parlava qualche volta della sua lotta in clandestinità, nella Resistenza, come staffetta partigiana con il nome di Rosario. Mi diceva che non aveva mai avuto timore per lei, da gran combattente, ma aveva avuto paura per la sorte dei suoi figli e dei suoi fratelli minori. Mi raccontava con passione ed entusiasmo della sua esperienza di responsabile dell'Ufficio lavoratrici del sindacato negli anni Cinquanta, agli albori del sindacato di Giulio Pastore. Aiutava le donne - lei, da donna che aveva avuto la possibilità di studiare e laurearsi - a riscattarsi dalla loro condizione, anche dando istruzioni sulla propria igiene personale. Si era battuta, da sindacalista prima e da politica dopo, per la parità salariale, contro la precarizzazione del lavoro femminile. Dobbiamo a donne come Alessandra Codazzi le conquiste che anche oggi stiamo compiendo. compiendo. Proprio adesso, in un tempo nel quale abbiamo tanta responsabilità di cambiamento, dalla transizione digitale a quella ecologica, alla necessità di politiche demografiche,

ma l'essenza stessa dell'umanità. Ritengo che questo nostro tempo sia simile al suo degli anni Cinquanta ed è uno di quei momenti che abbiamo il privilegio di vivere. Noi dovremmo essere all'altezza della

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, sono passate quasi due settimane da quando ho chiesto al ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli la convocazione di un tavolo tecnico per discutere dei gravi problemi che attanagliano la filiera della pera. A metà ottobre ho partecipato all'assemblea generale dei pericoltori emiliani, che si è tenuta a Mirandola, in provincia di Modena. L'evento, dal titolo «Dalla catastrofe al cambiamento per la rinascita del settore della pera», ha rappresentato un momento importantissimo per discutere con oltre 300 agricoltori della crisi che il settore sta attraversando e delle gravi problematiche derivanti dalle dalle gelate tardive del 2021 e dalle altre emergenze fitosanitarie e anche di mercato, che colpiscono soprattutto le drupacee e le pere. Nel corso dei lavori abbiamo discusso dei numeri della crisi frutticola che sta investendo l'Emilia Romagna e che non ha precedenti nella storia. Basti pensare che stringe nella morsa circa 20.000 aziende agricole, 60.000 lavoratori e un patrimonio di oltre 50.000 ettari complessivi di frutteti. Questo senza contare il valore economico dei settori della trasformazione, distribuzione e dell'indotto

mettono sotto scacco quasi il 70 per cento dell'intera produzione agricola regionale delle pere. Il grido d'allarme dei pericoltori italiani non va ignorato, perché quanto sta accadendo nel loro settore è lo specchio di quanto avviene in generale in tutto il settore ortofrutticolo, duramente colpito anche dalla pandemia. Conseguenzialmente, denuncio l'inerzia del Governo Draghi, già da molti mesi, ma vengo inascoltata. La filiera ortofrutticola, in questo caso il comparto delle pere emiliane, eccellenza italiana, non può assolutamente attendere ulteriormente risposte e aiuti. Il mio appello è anche quello degli imprenditori agricoli, ma al momento è rimasto lettera morta. Ora è il momento di agire. Il ministro Patuanelli dica finalmente da che parte stare, se da quella delle piccole e medie imprese agricole, cuore pulsante dell'agricoltura nazionale e del *made in Italy*, le cui proteste si fanno ogni giorno più vibranti, o se vuole continuare a stare dalla parte dei grandi gruppi del settore. Signor Presidente, Adelina Sejdini è la donna morta gettandosi da ponte Garibaldi lo scorso 6 novembre qui a Roma. Adelina Sejdini l'abbiamo conosciuta in parecchi in questa sede, perché venne a portare la sua testimonianza nel corso dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione in 1a Commissione e e venne nonostante le sue precarissime condizioni di salute, nonostante un tumore invasivo di tipo C3, nonostante la chemioterapia cui era sottoposta e nonostante la mastectomia bilaterale che aveva appena subito al momento della sua presenza qui. Venne perché - sono le sue parole «fino al mio ultimo respiro darò il mio contributo alla lotta alla tratta perché provengo da quello che definisco l'inferno della prostituzione». Chi era Adelina Sejdini non lo apprendiamo dai giornali, ma dalle sue vive parole e dalla sua testimonianza. «All'età di diciassette anni e mezzo venni sequestrata con la forza ed ero ancora come mia madre mi aveva fatto. Fui costretta a salire su una macchina e portata in un *bunker*, di quelli sotterranei che si usano nei Paesi in cui c'è la guerra, dove venni violentata da un gruppo di persone. Fatto questo, mi portarono poi in una casa, poi in un campeggio e mi hanno venduta di banda in banda con destinazione "prostituzione in Italia", dove sono arrivata a bordo di un gommone, sul quale c'erano tantissime altre ragazze. Prima di arrivare al gommone però, voglio ricordare il campeggio delle torture. In quel campeggio c'erano tantissime ragazze che venivano torturate e violentate, tutte destinate allo stesso gommone. Su quel gommone c'era anche la Polizia albanese che, dandoci pacche sulle spalle, ci raccomandava di fare tanti bei soldi al nostro arrivo in Italia. Io sono finita a prostituirmi nel Varesotto. Ho subito l'inferno delle torture e delle botte, tant'è che tutt'oggi porto le cicatrici sul mio corpo: ne ho una sulla gamba destra che mi hanno fatto aprendomi un taglio profondo con il coltello e mettendoci del sale dentro, per poi legarmi e farmi infine una doccia ghiacciata. La Polizia del Varesotto tutti i giorni veniva a chiedermi chi mi avesse messo lì e a dirmi che potevano aiutarmi, ma io avevo paura di fidarmi di loro perché associavo la loro divisa a quella della Polizia albanese. Un giorno, però, decisi di farlo, ribellandomi a un inferno di schiavitù e torture, ma lo feci solo dopo quattro anni. Grazie alla mia denuncia sono state liberate dieci ragazze, 40 sono stati gli arrestati, 80 i denunciati e tutti sono stati condannati a una pena dai quindici ai vent'anni di carcere. Così mi sono detta: visto che la vita è tanto bella, soprattutto se si è libere di scegliere e di fare quello che si vuole, allora tantissime altre ragazze potevano essere libere di scegliere. Ne ho, quindi, fatto una missione e, in collaborazione con le Forze dell'ordine, ne ho salvate numerose. La prostituzione sul nostro territorio - dico nostro anche se non sono nata in Italia, ma mi sento italiana e parte della società italiana - vede più di 120.000 donne vittime di tratta. Posso dirlo sia da *ex* vittima del *racket* della prostituzione sia da attivista. Bisogna fermare la domanda e rivolgo questa mia richiesta e questa supplica a chi ha il potere di fare qualcosa. Come fermare la domanda? Ad esempio, sanzionando i clienti. Per quanto riguarda la prostituzione sul territorio italiano, nessuna donna si può prostituire da sola, neanche se lo vuole. C'è chi parla di legalizzare i bordelli e le cosiddette zone rosse. Se oggi fossi ancora schiava, avrei paura che qualcuno mettesse una bomba a casa mia contro i miei familiari e io starei dentro a quel bordello. Così i miei sfruttatori prenderebbero i soldi, mentre lo Stato incasserebbe le tasse. Io, come qualsiasi altra donna, mi aspetto da chi rappresenta lo Stato - mi riferisco alle istituzioni, al Governo e a chi ha potere - di offrirmi opportunità dignitose. Io non tifo per alcun partito - lo giuro davanti a Dio - ma vi dico che modificare la cosiddetta legge Merlin eliminando il reato di favoreggiamento alla prostituzione vuol dire dare libertà alla criminalità organizzata. Infatti, se gli angeli in divisa così chiamo i poliziotti e, in generale, tutti gli appartenenti alle Forze dell'ordine - riescono ad avviare una prima indagine per inchiodare i delinquenti che sfruttano migliaia di ragazze è proprio grazie al reato di favoreggiamento della prostituzione. Quindi, dico un forte no all'apertura dei bordelli e all'abrogazione del reato di favoreggiamento della prostituzione. Concludo, Presidente Adelina dice ancora: «Mi rivolgo con forza a chi ha il potere di fare qualcosa per queste ragazze. Prostituirsi in Italia già non è reato. Che cosa si vuole legalizzare? La schiavitù? Chi vuole prostituirsi da danni può andare a pagare le tasse, ma non lo fa. In conclusione, giuro davanti a Dio che se sono qui oggi è per dirvi che personalmente ho subito tutti i tipi di torture e quelle che ho subito io le stanno subendo tutte le ragazze. Fate qualcosa per queste ragazze, non permettete che venga legalizzata la schiavitù della prostituzione e vengano aperti i bordelli. il mio medico mi dovesse dire che sto per morire e mi chiedesse di esprimere un ultimo desiderio, direi che il mio desiderio è fermare la domanda di prostituzione che genera la tratta di esseri umani. Non lo dico tanto per dire, ma lo penso veramente. Bisogna fermare la domanda con sanzioni ai clienti, perché sono consapevoli». Questo è l'appello di Adelina Sejdini.